L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo

*(PD)*. Signor Ministro, abbiamo oggi in Italia una grande occasione, quella di riformare davvero il sistema lavoro nella direzione delle politiche attive, sia nei percorsi di accesso che in quelli di ricollocazione. Con un tasso di disoccupazione giovanile così alto, è indispensabile che le nostre ragazze e i nostri ragazzi abbiano fiducia nelle istituzioni e nei servizi al lavoro quando cercano un'occupazione, per compiere un primo approccio al lavoro e non scoraggiarsi. Solo dalla creazione di occasioni e di opportunità si possono aprire le porte per la realizzazione personale in ambito lavorativo in maniera responsabile ed autonoma. Le chiedo allora, signor Ministro, l'andamento di Garanzia giovani, proprio nella direzione della fiducia dei giovani scoraggiati nell'avvicinarsi al sistema dei servizi offerti, e come d'altro canto ha risposto finora il sistema. In particolare, le chiedo di riferirci delle possibili sinergie tra Garanzia giovani e le altre politiche attive sviluppate dalle Regioni, ed ancora se ci sono dati sulla creazione d'impresa dei giovani. Analogamente, per le persone che perdono il lavoro, è interessante comprendere come si organizzerà il sistema dei servizi, soprattutto nella creazione di un'agenzia nazionale per l'occupazione, perché perché il contratto di ricollocazione, appena approvato nel decreto legislativo attuativo *jobs act*, sia occasione per realizzare il principio di condizionalità, rispetto alla disponibilità reale di trovare un altro lavoro e spostare il centro delle politiche del lavoro da quelle passive a quelle attive. Signor Ministro, premettendo che l'attuazione del *jobs* del *jobs* *act* mira all'abolizione, a partire dal 1° gennaio 2016, del contratto a progetto per ora solo nel settore privato, queste misure sono giustificate dalla volontà di eliminare il precariato e garantire maggiore stabilità ai lavoratori. Noi invece avremmo voluto preservare, perché adeguato al contesto economico ed occupazionale del nostro Paese, ciò che è stato realizzato attraverso la legge Biagi, come il co.co.pro., in grado di rendere flessibile il nostro mercato del lavoro e più agevole l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Considerato che dagli ultimi dati ISTAT, relativi al mese di febbraio, il tasso di disoccupazione è aumentato fino al 12,7 per cento, in crescita rispetto a gennaio; che un dato ancora più allarmante riguarda la disoccupazione giovanile, che sempre a febbraio raggiunge il 42,6

attuali contratti flessibili in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

a risolvere il problema occupazionale italiano. A mio avviso - e purtroppo non sono il solo a pensarla così, e poi ci sono anche i dati - avete intenzione di distruggere, una volta e per sempre, il nostro tessuto economico composto da piccole imprese e lavoratori, svendendolo all'estero, come avete fatto con la moneta. Vi contrasteremo. Ministro, tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 1 elenca principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, si chiede cosa ha in programma il Governo circa la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione per coloro i quali hanno minore probabilità di trovare occupazione, tenuto conto che l'unica cosa che avete fatto è togliere le agevolazioni strutturali per l'assunzione dei disoccupati di lunga durata, che erano previste dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407. Inoltre, con l'introduzione del nuovo contratto a tempo indeterminato, ma a rischi decrescenti - chiamiamolo nella sua sostanza - avete ulteriormente precarizzato l'Italia e, cosa ancora più grave, avete esteso la disciplina del licenziamento facile anche a quelli collettivi, fregandovene del parere che il Parlamento aveva espresso in Commissione lavoro. Ora, il comma 7 dell'articolo 1 delega il Governo a riordinare i contratti di lavoro vigenti. Anche qui sarà un massacro sociale, e già lo so.

siamo pertanto a sollecitarla in questa sede a che vi si dia piena attuazione, ovvero che tutte le deleghe che sono in esso descritte trovino attuazione attraverso gli opportuni decreti delegati.

avete la possibilità di ulteriori tre mesi, e quindi fino al 16 settembre, in relazione al momento di consegna alle Camere stesse. In modo specifico, però, voglio attirare la sua attenzione sull'esigenza di dare piena attuazione anche a deleghe, di cui forse si è parlato meno in questo periodo, quella relativa al salario minimo, che non solo è una tutela per segmenti di lavoratori oggi non protetti dalla contrattazione collettiva, ma è anche istituto utile a riformare la contrattazione collettiva, sospingendola quanto più nella sede aziendale o territoriale. Dall'altra parte, vi è il testo unico semplificato, ossia quello che dovrebbe riunire tutte le disposizioni sui rapporti di lavoro e sulle tipologie contrattuali. Fu il Presidente del Consiglio a parlare fin dall'inizio di un testo unico semplificato, traducibile in inglese. A questo proposito, ricordo che, per avere un testo unico traducibile in inglese, basta rifarsi strettamente alla regolazione comunitaria, che in inglese è già espressa.

*(Misto-SEL)*. Signor Ministro, come saprà, è da settimane ormai che i lavoratori della Fincantieri stanno scioperando in massa in tutti i cantieri italiani: difendono la democrazia con la lotta ed un lavoro dignitoso. In questi giorni, tutti abbiamo letto - quindi penso anche lei - dei *microchip* da inserire negli scarponi o nei caschetti dei lavoratori, della mezz'ora in più di lavoro gratis che dovrebbero fare e di delocalizzazioni. La notizia, qualora venisse confermata - e le chiedo lumi in merito - sarebbe grave, e paradossalmente ancora di più in quanto parliamo - lo ricordo - di un'azienda a partecipazione pubblica. Ricordo ancora che pochi giorni fa l'Europa ha bocciato severamente il controllo a distanza dei lavoratori. Per questo, signor Ministro, la invito e le chiedo di convocare da subito le parti, aziende e sindacati, anche perché sono a conoscenza del fatto che il sindacato ha già chiesto un incontro, ma non ha ancora ricevuto risposta. Credo che la lotta, quand'è democratica e dignitosa,

l'epoca dei vantaggi fiscali, il neoassunto è licenziabile: basta indennizzarlo con le famose due mensilità per ogni anno lavorato.

ci dicono che il programma Garanzia giovani vede oggi registrati 491.000 giovani, di cui 15.000 si sono registrati solo nell'ultima settimana.

enti che gestiscono i programmi, hanno avviato prima la parte strutturale di profilazione e di attivazione della relazione e poi hanno attivato le misure, che naturalmente sono partite mesi dopo, e quindi cominciano ad avere oggi una risposta. Consideriamo - ad esempio - che, all'interno di tali misure, c'è il servizio civile, che si sta sviluppando proprio in questo momento. Dal punto di vista degli elementi in nostro possesso, siamo in grado di dire che le Regioni, che avevano e che hanno in corso degli specifici programmi per la promozione della occupabilità dei giovani, hanno integrato questi progetti con il progetto Garanzia giovani. Abbiamo progetti in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna e in Toscana.

delle Regioni in questo senso, esse vengono normalmente coordinate tra il programma Garanzia giovani e il programma di attivazione delle Regioni. Per quanto riguarda la creazione di imprese da parte dei giovani, credo possa essere utile citare il dato secondo cui 17 Regioni

in generale, Garanzia giovani è stata anche un'occasione per portare i servizi per l'impiego a sviluppare un'azione che, storicamente, non avevano mai sviluppato. fare legittimamente delle osservazioni da questo punto di vista, ma 244.000 giovani che si sono presentati ai centri per l'impiego, che hanno avuto una profilazione e devono essere seguiti o assistiti, sono sicuramente un dato importante, in prospettiva futura. Noi abbiamo, cioè, qualcosa di prezioso in mano: una banca dati, un sistema relazionale, che è tutto materiale, sul quale bisogna lavorare. Quindi, abbiamo intenzione di sviluppare il lavoro dei centri per l'impiego potenziandoli, per poter gestire al meglio questo tipo di situazione in prospettiva futura.

gli interventi che abbiamo realizzato sul piano normativo e, contemporaneamente, sul piano della decontribuzione e sul piano fiscale, togliendo dalla base di calcolo IRAP il costo del lavoro da contratto di lavoro a tempo indeterminato, producano questo esito, cioè un significativo trasferimento da contratti a tempo determinato, da collaborazioni a progetto e da altre tipologie contrattuali a contratti a tempo indeterminato. il passaggio da contratti precari o da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato sia una cosa utile ed importante che doveva essere favorita. Naturalmente noi ci auguriamo anche che, oltre ad un trasferimento di contratti, ci siano nuovi contratti di lavoro aggiuntivi. La norma non produce nuovi contratti di lavoro - questo mi pare piuttosto ovvio - ma noi pensiamo che avere un contratto a tempo indeterminato metta le persone nella

precari e a tempo. Banalmente, è possibile ottenere un mutuo o fare una scelta che garantisca meglio o faccia immaginare meglio la propria prospettiva di vita. Questo dovrebbe migliorare anche le condizioni dei consumi interni del nostro Paese ed essere uno degli elementi che, insieme agli altri, può produrre un miglioramento generale.

nostro parere - l'apertura del mercato del lavoro, per tutto quanto ho appena finito di dire, rappresenta un'opportunità anche per le persone che sono disoccupate da più lungo periodo. poi messo in campo un'azione, che è quella che stiamo predisponendo per i nuovi decreti, che riguarda le politiche attive ed il riordino degli incentivi. È vero che c'è stata la soppressione di una tipologia di intervento precedente, ma oggi pensiamo di abbinare la presa in carico attraverso i contratti di ricollocazione ed uno specifico incentivo, perché la somma di queste due azioni e il cambiamento strutturale della tipologia di contratto

dei pareri delle Commissioni, il Governo ha sempre agito e ha intenzione di agire in conformità con le previsioni normative, e naturalmente si assume la responsabilità delle decisioni che adotterà. Utilizzerà e valuterà i pareri delle Commissioni, come la legge propone, e, sulla base delle proprie valutazioni, li utilizzerà nelle sue decisioni finali. Rispetto alla scelta che andrà a fare, naturalmente sarà valutato e considerato dalla pubblica opinione, così come dagli stessi parlamentari. Per quanto

vista, lo stato delle situazioni è noto. Noi siamo intenzionati a procedere, secondo i tempi, a completare questa delega per la parte che fa riferimento al tema

Qualora e laddove ci sia un'esigenza di un intervento del Governo, questo è pronto a intervenire perché tutto ciò che è previsto sia rispettato.

Sono soddisfatta perché per il Governo è anche un'occasione - come ha detto il Ministro - per fornire all'Italia un sistema vero di politiche attive e di servizi al lavoro efficienti. Ci auspichiamo che quanto prima ci sia il decreto attuativo del *jobs act* sulle politiche attive e sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego, che potrà mettere a sistema tutto e potrà davvero intervenire per le esigenze dei giovani che cercano lavoro e per chi lo perde con i contratti di collocazione, come ricordavo prima. XVII)*. Signor Ministro, apprezzo il suo ottimismo e il suo ben pensare ma, per le condizioni economiche del Paese, devo ribadire che la flessibilità introdotta dalla legge Biagi soddisfaceva contemporaneamente due esigenze che ancora oggi sussistono. In primo luogo, dava alle imprese uno strumento in grado di sopportare i costi aziendali adeguandoli alle *performance* produttive e, in secondo luogo, favoriva l'occupazione e l'accesso ai giovani nel mondo del lavoro. Non c'è un pregiudizio contrario alla stabilità, ma è un principio che, stando così le cose, non può essere realizzato facilmente. Pertanto, la scelta più opportuna sarebbe stata quella di mantenere i contratti flessibili.

È ovvio che, se io trasformo, attraverso il *jobs act*, il contratto a tempo indeterminato in contratto ormai senza più tutele, a rischi decrescenti, lo stesso

ossia il nuovo statuto dei lavoratori. Lo statuto dei lavoratori è stato già modificato in alcuni contenuti fondamentali, ma il disegno di legge vi dà la possibilità di sostituirlo con un testo unico innovativo, non meramente compilativo (cioè di norme vigenti), combinandolo anche con le deleghe alla semplificazione, ma tale da darci un impianto regolatorio semplice, certo, speriamo certamente applicato,

Se le parti avessero trovato un accordo, non staremmo qui a parlare. Sono settimane che i lavoratori stanno scioperando. La invito, quindi, di nuovo, a convocare le parti, perché credo che il Governo debba assumersi questa responsabilità. In caso contrario, qui parliamo di aria fritta. E io non sono capace di parlare di aria fritta, ma di fatti concreti.

di pochissima efficacia. È vero che c'è stata una piccola ripresa, ma è dipesa da fattori esterni. Per esempio, le manovre della BCE hanno consentito di avere denaro a bassissimo prezzo e, pertanto, il costo del nostro debito è pressoché nullo; il cambio tra dollaro ed euro è favorevolissimo per chi esporta;

potrà, nella seconda tornata di risposte, tornare sull'ultimo punto della domanda della senatrice Parente riguardante il nesso tra tra contratto di ricollocazione e condizionalità, che penso sia molto importante sul terreno della ristrutturazione dei servizi per l'impiego. La domanda relativa, invece, alla materia previdenziale è la seguente. Noi siamo arrivati, purtroppo, purtroppo, soltanto nel 2011, con due decadi di ritardo rispetto al tempo che sarebbe stato necessario, ai provvedimenti indispensabili per il riequilibrio finanziario del nostro sistema pensionistico. Questo ha reso necessario fare le cose in un tempo rapidissimo e senza quella gradualità che avrebbe consentito di mettere in atto le misure che,

mi chiedo se, di fronte al problema di chi ha cinquanta-sessant'anni ed ha maggiore difficoltà a trovare una nuova occupazione di quanto non abbiano le persone in età più giovane, la soluzione non debba consistere nel prevedere un'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione legata a misure, appunto, di promozione dell'*active ageing*. Questo, naturalmente, è del tutto alternativo rispetto a quanto è chiesto da altre parti politiche, cioè di tornare indietro rispetto alla riforma del 2011. Su questo punto, però, credo che il Governo debba mettere in campo una progettualità che ancora non si è compiutamente espressa e chiedo, in proposito, l'orientamento del Ministro e del Governo.

se da una parte hanno aumentato la sostenibilità fiscale del sistema pensionistico italiano nel lungo periodo, dall'altra hanno introdotto parametri di grande rigidità, fortemente penalizzanti in particolare per i lavoratori più anziani, che hanno visto allontanarsi la prospettiva della pensione. Considerato che il sistema, pur se economicamente sostenibile e caratterizzato da forti disomogeneità e squilibri generazionali, con lavoratori costretti a continuare la propria attività

mesi e non più prorogabile. In particolare, chiediamo se sia concretamente configurabile un meccanismo di anticipazione della pensione per chi perde il lavoro ed è prossimo alla pensione, anche considerando l'opposizione dell'Unione europea sul tema specifico. quanti lavoratori esodati devono essere tutelati ancora, dopo sei interventi che hanno coinvolto circa 170.000 persone, a fronte di una spesa di oltre 11 miliardi di euro.

Questa tipologia di lavoratori - oltre 400.000 - avrà, a causa delle vostre scelte, ulteriore instabilità e precarietà; precarietà che questo Governo ha accentuato con il *jobs act*. I lavoratori stagionali non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno,

introdotto nella legge di stabilità, per poi sospendere il lavoratore per sei mesi, negandogli anche di beneficiare dei tre mesi di NASPI. Questa sarebbe una cosa gravissima. Ministro, lei stesso ha dichiarato anche prima che con la riforma del lavoro non si crea lavoro, ma ha omesso di dire di aver tolto ai lavoratori diritti e forme di garanzia economica: forma di garanzia del reddito che noi del Movimento 5 Stelle stiamo portando avanti con forza in Commissione lavoro attraverso la nostra proposta di reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura attiva e universale di vera tutela del cittadino, di equità e giustizia sociale. Ciò adeguerebbe veramente l'Italia ai modelli di flessibilità e sicurezza dei principali Ministro, fuori da queste Aule c'è un grande bisogno di risposte certe e chiare. Nove milioni di cittadini vivono in precarietà e gravi difficoltà quotidiane. Ministro, chiedo che questo Governo prenda una posizione netta e chiara davanti agli italiani sulla nostra proposta di reddito di cittadinanza e chiedo inoltre cosa intende fare per risolvere il grave, gravissimo, problema dei lavoratori

le conseguenze. Intende completarla, con particolare riferimento alla ricongiunzione senza oneri di tutti i periodi contributivi, perché non un euro accantonato debba essere disperso? flessibilità di età di uscita su base contributiva (proprio perché prendo in base a quanto ho versato); versamenti volontari del datore di lavoro oltre che del lavoratore, anche oltre il periodo lavorato in modo da poter coprire quanto più i periodi di non lavoro in un tempo nel quale la discontinuità lavorativa può, purtroppo, essere frequente; possibilità di versamenti volontari per recupero di periodi di studio quanto più modulati, non a taglia unica, nella logica contributiva (più verso e più avrò); avrò); incentivi per questi versamenti che siano ancor più incoraggianti all'afflusso di risparmio previdenziale anche al cosiddetto primo pilastro di previdenza obbligatoria; obbligatoria; complementarietà fra i pilastri, fra quello obbligatorio e i due volontari, quello collettivo e quello individuale, in modo tale che sia sempre possibile, a certe condizioni irrobustire innanzitutto la prima pensione, la prima pensione, quella fondamentale, anche traslando risorse dai due pilastri a carattere volontario a quello a carattere obbligatorio. *(Misto)*. Signor Ministro, in considerazione del fatto che annualmente viene allungato il requisito anagrafico, ai fini del calcolo dell'età pensionabile, di tre mesi più o meno in linea con la politica europea, in virtù dell'allungamento della speranza di vita, ritengo sia necessario avviare una seria riflessione sul tema. Se da un lato si vive più a lungo, altrettanto vero è che la qualità della vita è peggiorata

se non occorra mettere in quiescenza i lavoratori ad un età congrua rispetto al ruolo ricoperto, ovvero rivedere anche tutta una serie di lavori usuranti, i quali non possono essere catalogati solo in funzione delle ore, come ad esempio chi svolge lavoro notturno:

Occorre garantire il lavoro, quello di qualità però. Ciò è possibile soprattutto attraverso un sano ricambio generazionale. In altri termini, ciò è fattibile operando un automatico aggiornamento delle capacità lavorative, ossia al passo col tempo. Inoltre, per garantire un ricambio generazionale occorrono politiche di *welfare* migliori. Ricordo, infatti, che ad oggi le donne, in termini percentuali, vengono occupate meno degli uomini, anche in virtù del fatto che le stesse debbono far fronte a più lavori: al lavoro che svolgono, se ce l'hanno, oltre al carico familiare (cura dei figli e assistenza

MpA, NPSI, PpI, IdV))*. Signor Ministro, piangere lacrime di coccodrillo è un modo di dire di uso comune in Italia e si riferisce a chi finge di provare dispiacere quando in realtà è disinteressato o peggio, compiaciuto, rispetto al fatto che causa dolore a qualcuno. Il detto trae origine dal mito secondo cui i coccodrilli verserebbero lacrime di pentimento dopo aver ucciso le loro prede e averle divorate. Così, l'ex ministro del lavoro Fornero, con la sua riforma del sistema previdenziale, dopo aver divorato l'aspettativa previdenziale di milioni di lavoratori italiani che non sono più potuti andare in pensione e dopo aver così

noi abbiamo bisogno che i nostri figli siano attivi, che siano i giovani a trovare lavoro, soprattutto nella sanità, nella ricerca, nella scuola, nella pubblica amministrazione, nel settore manifatturiero, dove ci sono le eccellenze italiane. Se

roghi e di streghe, non sono più adatti a questi tempi. Abbiamo bisogno di queste forze per rilanciare lo sviluppo in Italia, né più né meno di quello che è successo nel 1984, quando ministro del lavoro era De Michelis e presidente del Consiglio

Da parte nostra, signor Ministro, reputiamo che i ricorsi saranno inevitabili, perché c'è una disparità di trattamento inevitabile e forse c'è anche una violazione del principio costituzionale

Come ha correttamente affermato l'interrogante, le assunzioni a tempo indeterminato, esclusa la pubblica amministrazione e il lavoro domestico, nel primo bimestre del 2015 sono state 79.000 in più rispetto allo stesso periodo 2014. Si tratta quindi, in sostanza, di una differenza tra il numero assoluto

altri numeri non possiamo fare delle valutazioni perché il sistema non rileva le situazioni di contratto o di lavoro autonomo:

le condizioni alle quali si offre il nuovo posto di lavoro ed il vincolo «in termini di obbligo»: è chiaro che, se non sarà così, questo meccanismo tendenzialmente non funzionerà. Il tema della condizionalità è dunque assolutamente essenziale.

riferimento a che cosa si pensa di fare. Noi pensiamo che sia necessario rimettere mano a questa situazione, perché effettivamente - non esprimo - non esprimo qui considerazioni puntuali rispetto alla riforma - oggi verifichiamo l'esigenza di cambiare una serie di situazioni. In particolare, abbiamo un problema di tipo sociale evidente: i lavoratori che arrivano vicino alla maturazione del requisito di pensionamento, ma che non sono più coperti da ammortizzatori sociali, rischiano di trovarsi in una terra di nessuno e di questo occorre tener conto. Da una parte abbiamo cercato di affrontare affrontare questo tema utilizzando l'ASDI, l'assegno di disoccupazione, cercando di prolungare questo istituto, ma il problema rimane, per cui dovremo trovare la maniera di affrontarlo.

quantificare e qualificare le risorse che saranno necessarie per gestire le scelte che andremo a fare eventualmente in quella sede. Oggi dunque

riferimento. Quindi abbiamo un tema sociale, quello che dicevo, ed abbiamo un tema generale di flessibilità in uscita. Questo è l'altro elemento sul quale ci stiamo esercitando, cioè valutare quali possono essere le modalità attraverso le quali produrre questa situazione. A questo è collegata la problematica che avete proposto: chiamiamola staffetta generazionale o come vogliamo, abbiamo comunque un tema di connessione tra

rispetto ai giovani, cioè rispetto alle persone che non avevano un'opportunità di lavoro. Non voglio fare ora una traslazione scorretta, però il tema che ci proponeva il senatore Ichino in termini di come gestire una fase di uscita dal mercato del lavoro o dalla propria professione in maniera graduale e sostenibile, sia sul piano previdenziale che sul piano personale, parla di entrambe le questioni che sono state qui citate. Insieme a questo naturalmente abbiamo i temi che il senatore Sacconi ci ha proposto. Io credo che questi debbano essere ricompresi nella riflessione che andiamo a fare, perché essi in qualche modo aiuterebbero

intervenire rispetto a questo tipo di situazione. Queste sono tematiche che affronteremo all'interno di questa vicenda. C'è poi un altro tema, che è stato proposto dal senatore Divina e che riguarda la disparità di trattamento proposto dal senatore Divina e che riguarda la disparità di trattamento sulle penalizzazioni, cioè la scelta fatta dalla legge di stabilità. In questo momento il Governo non ha in previsione

Questa finalità chiaramente non è perseguibile rispetto alle persone che sono già in pensione; quindi non si coglierebbe questo obiettivo. Esiste il tema di una diversità di condizione che si va a determinare, ma, sul piano generale, credo che normalmente o molto spesso, quando si fa un intervento su una situazione di fatto, si produce sempre una situazione di prima e di dopo e quindi non si risolve questo tipo di problema.

prevede una prestazione collegata alla pregressa storia contributiva di ogni lavoratore. Questo è un tema che certamente riguarda i lavoratori stagionali, ma riguarda anche i lavoratori in generale. Quella norma,

nell'andamento a regime di questa norma; in ogni caso, riteniamo che sia necessario trovare una modalità che consenta alle persone che si troveranno in questa situazione di avere davanti un lasso di tempo in forza del quale sanno quello che accadrà e si attiveranno

Mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta del Ministro, sia per il completamento della risposta alla domanda presentata dalla senatrice Parenti, sia per la parte relativa all'invecchiamento attivo e all'impegno del Governo su questo che credo debba diventare un nuovo capitolo molto importante della nostra politica del *welfare*. *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, purtroppo l'approccio del Governo su una riforma così delicata mi sembra ancora essere vago e un po' approssimativo. Devono essere trovate soluzioni che garantiscano ai lavoratori maturi di poter andare in pensione ad una età ragionevole e prestabilita, in una staffetta generazionale per i giovani che subentrano nel mondo del lavoro ai più anziani. però, le pesanti penalizzazioni sulla previdenza complementare, che il Governo ha introdotto con l'ultima legge di stabilità, dimostrano scarsa lungimiranza e incomprensione della realtà, e non ci fanno ben sperare per il futuro. Ministro, lei mi sta dicendo in poche parole - annuncia, annuncia - che forse farete qualcosa, ora si vedrà. Il problema è che i lavoratori stagionali sono veramente molto preoccupati. I vostri annunci solo soltanto propagandistici e basta: mi dispiace annunciare questo. I dati confermano ciò che io dico. Ministro, la verità è che in febbraio si sono registrati 44.000 occupati in meno e 23.000 licenziamenti in più, nonostante i vostri *tweet* e annunci. La disoccupazione oggi è al 12,7 quindi, non sono per niente soddisfatta di questa sua risposta, e non sono solo io a manifestare insoddisfazione ma parlano i numeri, i fatti e gli italiani. Ministro, sono sicura che i lavoratori stagionali sarebbero felici di sentire la sua risposta direttamente martedì, durante la manifestazione. Se vuole, magari, ci andiamo insieme.

del lavoro, sostitutivo dello statuto dei lavoratori; e poi perché, con riferimento al completamento della riforma previdenziale e al compimento della logica contributiva, ha condiviso l'esigenza di procedere ad una serie di decisioni. Non ce ne ha dato dettaglio, ed era giusto che così fosse in questo momento, anche perché ogni qual volta parliamo di pensioni il Governo è tenuto a far di conto nel breve e nel lungo periodo, ma mi sembra di poter cogliere nella sua risposta che, a differenza di quella riforma Fornero, oggi pensiamo a numeri, ma anche a persone. Guai se pensassimo solo ai numeri e non anche alle persone. non sono così soddisfatta, direi, in quanto alla fine non ci è stata data una risposta vera e propria per quanto riguarda il sistema pensionistico. Si continua, appunto, a perorare la causa e a chiedere di rivedere le norme sulle pensioni. Ci siamo anche affidati al nuovo presidente INPS Boeri, il quale deve fare un conteggio che poi ci dirà, e si spera che il Parlamento, insieme al Governo, produca qualcosa che dia una risposta effettiva alle persone. Mi sembra che oggi davanti al vostro Ministero c'erano di nuovo gli esodati che chiedevano di essere reintegrati in un sistema pensionistico. La legge Fornero ha prodotto un numero di esodati importante e li ha lasciati in un vuoto economico immenso.

un nuovo mondo lavorativo. È inutile che si faccia il *jobs* *act* e che si creino posti di lavoro attraverso sgravi fiscali, che potranno andare anche bene. Di fatto, però, è necessario liberare posti di lavoro, fare politiche in cui si implementa

Ma quale staffetta generazionale? Ci vuole un contratto, un patto generazionale di entrata e di uscita, ce n'è bisogno per lo sviluppo. La dose è questa:

Signor Ministro, è stato cortese, peccato però che le opinioni che abbiamo rimangano: forse il nodo è che l'abitudine di questo Paese e di questo sistema parlamentare è legiferare sull'onda delle emergenze.

La seduta è tolta